di un esame di abilitazione ad una professione. Penso quindi che si debba impostare l'attività di valutazione degli elaborati in maniera chiara, semplice e trasparente.

regole precise, sotto un duplice punto di vista. Il primo aspetto è quello della trasparenza, della chiarezza. Il candidato ha diritto a capire immediatamente, senza

«mediante una sintetica esposizione delle ragioni e dei presupposti della valutazione o, in alternativa,» - ancora meglio - «annotando osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato». Penso che questo emendamento sia fondato sulla ragionevolezza

"in una prova scritta avente ad oggetto la redazione di un atto che postuli la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale in materia di diritto e procedura civile o di diritto e procedura penale o di diritto e giustizia amministrativa".

fa cogliere se si tratta di giurisprudenza affastellata o criticamente utilizzata.

anche il cercare tra le diverse massime giurisprudenziali quella che più attiene al caso concreto è dimostrazione della validità del tirocinio. Se il problema è quello di leggere e correggere con più difficoltà i testi degli elaborati prodotti dai giovani, una una correzione attenta fa apprezzare e valutare la formazione del giovane così come è avvenuta nel corso di due anni e mezzo

46.212 e 46.218.

dovrebbe leggersi così: «I costi per l'espletamento delle procedure di esame devono essere posti a carico dei soggetti partecipanti».

«è tuttavia consentito l'ausilio del testo di legge con i soli giurisprudenziali»: manca una parola, anche se il concetto è chiaro. Qui vi è un problema di fondo, perché le osservazioni del senatore Li Gotti sono senz'altro pregevoli.

non sia previsto l'uso dei codici commentati con la giurisprudenza. Si risponde giustamente che lo studio della giurisprudenza deve essere un fondamento di quello che si sta per fare, con un parere o con un atto di appello, ma non può essere sentito e usato come una forca caudina da parte di un soggetto che aspira, in questo caso, a superare un esame.

Qual è la ragione per cui si dovrebbe introdurre o continuare a mantenere l'uso di codici commentati con la giurisprudenza e ancora avere in disprezzo, in fin dei conti, l'uso della dottrina? È ovvio che abbiamo strumenti precisi cui far riferimento. Per esempio, nella redazione delle sentenze - a proposito di comunione tra la dottrina, la giurisprudenza e il foro - vi è il divieto di citare la dottrina: si può, cioè, citare la dottrina, con molta cautela, ma non la fonte della dottrina. A questo punto, bisogna evitare che i giovani, che hanno seguito un percorso formativo molto importante, abbiano l'istinto naturale di dire: «Beh, se io trovo una sentenza delle sezioni unite, a quella mi aggrappo come ad una boa di sicurezza». Credo che l'emendamento 46.900/4, pur avendo delle ragioni, debba essere respinto.

Commissione, che testualmente recita: «Il titolo di abilitazione alla professione di avvocato non attribuisce punteggio per i concorsi pubblici». Posso forse comprendere in parte la *ratio* della norma,

che è stata fatta a seguito del parere della 5a Commissione permanente. Ancora una volta mi sembra - e uso questa espressione quasi in chiave eufemistica - che ci troviamo di fronte ad un atteggiamento punitivo

alla luce delle norme in materia di contabilità e in generale di quelle di competenza della 5a Commissione. Pur trattandosi di una

per l'accesso alla professione forense. La formulazione che proponiamo si differenzia rispetto a quella del disegno di legge in alcuni punti, a nostro modo di vedere importanti e fondamentali in chiave di interpretazione generale del sistema. Attiro l'attenzione dell'Aula su alcuni di questi punti che, ripeto, ci sembrano importanti. Al comma 1, dove si fa riferimento al decreto del Ministro che nomina la commissione per l'accesso alla professione forense, suggeriamo che lo stesso decreto preveda modalità che garantiscano la terzietà dei commissari, l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità. Non dovrebbe essere necessario sprecare troppe parole per spiegare l'importanza di una disposizione di questo genere, che indichi ed attribuisca al Ministro la facoltà e il dovere di indicare di volta in volta i criteri che rendano funzionante e giusto il concorso o, per essere più precisi, l'esame per l'accesso alla professione forense. Non dovrebbero esservi difficoltà a votare una norma così concepita, che integra ed arricchisce il quadro di riferimento normativo. Nella stessa prospettiva, ancorché con riferimento ad un altro aspetto, si colloca l'indicazione del comma 5

5. Gli avvocati componenti della commissione non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine, né alla carica di rappresentante della Cassa nazionale di previdenza e assistenza nel turno elettorale immediatamente successivo all'incarico ricoperto, laddove il comma 6 della normativa contenuta nel disegno di legge prevede una fattispecie di ineleggibilità: non vieta cioè la candidabilità, e non evita quindi il rischio che possano verificarsi di fatto indebite commistioni tra l'esercizio delle funzioni di membro della commissione e una attività di propaganda politico associativa, ciò che per l'appunto si vorrebbe e si dovrebbe evitare. Per queste ed altre ragioni, su cui non mi soffermo perché risultano chiare dal testo del disegno di legge, riteniamo che l'emendamento in esame debba essere approvato dall'Assemblea.

L'articolo 47, al comma 1, prevede la composizione della commissione di esame per l'accesso alla professione forense. Fra le varie categorie dei soggetti che compongono la commissione, vi sono - come è sempre stato e come è fisiologico che sia - i magistrati. La norma, indicata nel disegno di legge, che sono componenti della commissione magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello; sostanzialmente, come è adesso e come è giusto che sia, magistrati di una certa esperienza, operativi nel giudiziario, con la percezione cioè dello stato vivo della giurisprudenza: magistrati che fanno i magistrati. È inevitabile che sia così; è inevitabile che un apporto - che definirei fondamentale - alla utile ed efficace selezione dei giovani avvocati sia dato dai magistrati che fanno i magistrati,

le parole che fanno riferimento alla qualifica di magistrato di corte d'appello e, quindi, di magistrato in servizio, e si precisa che i soli magistrati che possono far parte della commissione per gli esami di avvocato sono i magistrati in pensione. in pensione. Invito anche il Governo a rivedere il suo punto di vista su questo emendamento, perché è veramente assurdo. Il magistrato in pensione, nel migliore dei casi, è un magistrato in pensione da poco tempo e, sempre nel migliore dei casi,

Ricordo personalmente, quando ho presieduto la commissione d'esame nel distretto della corte d'appello di Venezia, che un noto magistrato, nominato come membro supplente della commissione - oggi presente in quest'Aula come senatore - non si presentò mai,

Carofiglio che la Commissione, soprattutto nella fase in cui si era costituito il Comitato ristretto, ha interloquito con varie aree degli operatori di giustizia

quanto emerge una sorta di incompatibilità sostanziale rispetto ai gravosi impegni che caratterizzano l'attività del magistrato. Oggi il senatore Longo ha fornito un esempio evidente rammentando come un autorevole magistrato qual è il senatore Casson non ha mai potuto partecipare ai lavori della commissione perché altri e più cogenti impegni lo obbligavano ad essere altrove. Dunque, abbiamo tentato di trovare una sintesi e di armonizzare il

Come Sottosegretario con delega devo continuamente autorizzare sostituzioni per magistrati impegnati nei processi. Spesso si disquisisce

che noi riteniamo utile e necessaria e, dall'altro, si viene incontro alle esigenze di una giustizia, allo stato, in difficoltà per l'ingente numero di cause ancora pendenti, che costituiscono un arretrato pesante

presiedere la commissione. D'altra parte, non è giustificabile il fatto che il magistrato in attività sia impegnato al punto tale da non poter presiedere una commissione che si riunisce ogni due anni, mentre il professore universitario e il ricercatore non sarebbero, impegnati allo stesso modo. non sono stato bravo a spiegare il concetto. L'idea che voglio precisare con estrema chiarezza è la seguente: in maniera categorica, attraverso l'indicazione tassativa dei soli magistrati in pensione, quelli in servizio è sbagliato. La possibilità, da conseguire eventualmente con una riformulazione che affido alla valutazione del relatore,

d'accordo con il senatore Longo

nomini gli ispettori che possono partecipare alle prove d'esame piombandovi in qualsiasi momento. Non si comprende perché vi sia questo inserimento improvviso del CNF nell'ambito dello svolgimento del concorso per praticanti avvocati.

è stato pubblicato - ed è tuttora *on line* - un articolo di Gaetano Basso e Michele Pellizzari in cui si dà conto di una ricerca econometrica

produce una correlazione molto forte, statisticamente rilevante, tra la giovane con un avvocato e la probabilità di accesso all'albo, alla professione. Ne risulta

Il nostro voto contrario su questo articolo, come sull'insieme dell'impianto di questa disciplina della materia nasce dalla consapevolezza che oggi sarebbe necessario riformare profondamente questo assetto, per garantire una effettiva mobilità sociale e una vera parità per tutti i cittadini nell'accesso alla professione forense. Lo stesso discorso potrebbe valere per la professione di notaio, dove pure si osserva e si studia la stessa stretta correlazione tra l'appartenenza familiare e la probabilità di accesso alla professione. Stiamo consolidando un sistema familista e corporativo, nel quale i legami familiari prevalgono sui criteri di merito. Questo è un errore che non ha effetti negativi soltanto sul piano dell'equità sociale, ma anche su quello dell'efficienza del nostro sistema-Paese.

conforme al relatore.

la disciplina precedente per l'effettuazione degli esami per l'accesso alla professione forense, per ragioni francamente di difficile comprensione. Noi riteniamo che, nel momento in cui si disciplina la situazione transitoria per l'esame, sia necessario creare una sorta di scivolo, di passaggio da una normativa all'altra e che quindi sia necessario indicare, nei termini che non

mi limito solo ad alcune sintetiche considerazioni. Il testo attuale prevede l'istituzione di un organo istruttorio e di uno decisorio. Mantiene la competenza in appello del Consiglio nazionale forense ed il ricorso in Cassazione. Ora, occorre portare a più avanzata evoluzione verso la terzietà e l'efficacia il sistema disciplinare che deve essere, sia nella fase istruttoria sia nella fase decisoria, terzo rispetto all'incolpato e quindi composto da soggetti non appartenenti al suo ordine territoriale e possibilmente, anzi interamente, esterno al sistema ordinistico.

deve mutuare tutte le regole dal giudizio ordinario per assicurare un giusto processo e quindi una decisione che sia adottata secondo principi costituzionali. Uno di questi è la terzietà del giudice oltre che, naturalmente, la possibilità di

anche il procedimento disciplinare per gli avvocati ai princìpi del giusto processo e il giudice degli avvocati alla terzietà ed imparzialità, che costituiscono ormai le fondamenta di qualsiasi

quindi operata una ricognizione a tutto campo delle esigenze più avvertite da parte degli ordini italiani: dai grandi ordini delle grandi città ai piccoli ordini di provincia.

ciò che l'avvocatura, in tutte le sue articolazioni, aveva voluto nei termini che sono stati scritti. La ragione per la quale i pareri che esprimerò saranno

*(PD)*. In realtà, gran parte degli argomenti sono stati già sviluppati sinteticamente ma efficacemente, in sede di illustrazione dell'articolo. Vorrei aggiungere qualcosa per collocare sistematicamente la nostra riflessione su questa norma. Si discute in questi anni di Consiglio superiore della magistratura e dunque della necessità, della opportunità di scorporare dalle funzioni del Consiglio superiore della magistratura la funzione giudicante e disciplinare. Si dice - e io sono d'accordo, fermo restando che bisognerà riflettere sulle modalità che è necessario costituire una Corte di giustizia per la responsabilità disciplinare di tutti i magistrati. Ripeto che sono d'accordo. Sarà un passo nella direzione di un Paese più moderno dal punto di vista del funzionamento delle sue istituzioni,

Se questo è corretto, se la quasi totalità di coloro che sono in questa Aula, indipendentemente dalla loro appartenenza alla maggioranza o all'opposizione, sono d'accordo sul fatto che la responsabilità disciplinare dei magistrati debba essere giudicata da un soggetto diverso da quello che ne amministra le carriere, ebbene, risulta davvero incomprensibile - non so se questo aggettivo si può utilizzare e non è troppo forte - una ridefinizione, in un passaggio epocale qual è quello della ricostituzione del quadro normativo della professione forense, delle regole per il processo disciplinare che mantenga, così come era in un passato remoto ed in un quadro istituzionale diversissimo, quella commistione inaccettabile che esiste tra chi definisce le regole, chi amministra e chi fa giustizia: perché quella disciplinare è una forma di giustizia. Questo è il motivo per cui noi sollecitiamo al voto favorevole su questo emendamento, e chiediamo la votazione

Il nostro emendamento ora in esame mira ad inserire nell'emendamento della Commissione il riferimento, nella individuazione delle ipotesi di incompatibilità, anche ai membri del Consiglio dell'ordine. Do lettura del testo dell'emendamento «Nell'ipotesi in cui l'indagato, l'incolpato, la persona offesa o danneggiata sia uno dei componenti del Consiglio istruttore di disciplina o del Collegio giudicante di disciplina, nonché in ogni altro caso di incompatibilità,

giudichi la stessa entità amministrativo-giudiziaria di cui fa parte il membro del Consiglio dell'ordine? Non vi è, chiaramente, la la medesima ragione che induce allo spostamento di competenza nel caso dei magistrati, o che induce allo spostamento di competenza ai sensi di questo emendamento 51.200 (testo Attiro l'attenzione della maggioranza perché, su una cosa di questo genere, che ha a che fare con il minimo dell'architettura e degli equilibri delle compatibilità, voti assieme a noi, e si voti tutti quanti assieme, accettando questo emendamento. In ogni caso, chiediamo la votazione

nei confronti degli avvocati vengano annotate, mediante una sintesi dei provvedimenti relativi, comprensiva di cause e motivazioni, negli albi circondariali e siano liberamente consultabili consultabili sui siti *web* degli ordini e del Consiglio nazionale forense. Sui medesimi siti *web* deve, inoltre, essere liberamente consultabile anche il provvedimento integrale. Quindi, se sono stati assunti provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni avvocati, riteniamo utile che questi siano messi

Mi auguro che almeno gli stenografi possano ascoltare. Signor Presidente, colleghi,

del vice ministro Vegas: ci auguriamo che il prossimo Consiglio dei ministri formalizzi questa scelta. Occorre anche un altro commissario dimissionario. Tuttavia il presidente vicario, tal Vittorio Conti, ex direttore centrale di Banca Intesa, continua a minacciare e ricattare i parlamentari, colpevoli di fare troppe interrogazioni sull'operato di un sepolcro imbiancato come la CONSOB, adusa ad adottare decisioni arbitrarie a danno dei risparmiatori e della povera gente, favorendo gli esclusivi interessi dei banchieri. Si dice: "cane non morde cane". Già a metà luglio, a seguito di un'interrogazione presentata sulla «parentopoli» CONSOB, ossia un sistema di assunzioni clientelari per chiamata diretta successivamente stabilizzate con concorsi interni (un vero e proprio scandalo che mi venne segnalato con un plico con tanto di firme e di indirizzi), questo burocrate, il signor Conti, con sicumera da veggente, da baraccone, affermò che il sottoscritto aveva presentato l'atto di sindacato ispettivo sulla scorta di un esposto anonimo. Quell'esposto non era anonimo, lo ribadii in Aula, dove richiamai l'attenzione della Presidenza del Senato

pubblicata da un quotidiano, questi burocrati della CONSOB hanno affermato testualmente che il senatore Lannutti fa troppe interrogazioni parlamentari, per le quali sono costretti a fare ricorso in cassazione su una sanzione

giacché mi so difendere bene, ma per le funzioni di un parlamentare, garantite dalla Costituzione.

mi so difendere e mi faccio valere, quindi non lo chiedo per me ma per la dignità di quest'Aula. Comunque, le rendo noto, signor Presidente, che di questo episodio ho già informato con una lettera sia la Presidenza del Senato, quindi il presidente Schifani, il Presidente della Corte costituzionale, sia il Presidente della Repubblica. Questi signori delle Autorità non possono permettersi di minacciare e ricattare un parlamentare nell'ambito delle sue funzioni. *(Applausi

ma nessuno può interferire nel diritto-dovere di qualsiasi parlamentare di qualsiasi Gruppo politico di svolgere la sua funzione e la sua attività, attività, di cui è parte sacrosanta il sindacato ispettivo. Da questo punto di vista, lei ha certamente la solidarietà dell'intero Senato, perché nessuno può dire a un parlamentare se deve presentare o non presentare interrogazioni o altri strumenti propri della sua attività,

di cittadini non italiani che spesso sono in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno e che si sono autodenunciati, assumendosi la responsabilità di intraprendere un'iniziativa politica chiedendo la regolarizzazione. Ebbene, alcuni di questi sono stati fermati

in questi giorni è in discussione l'Atto Senato n. 2322, meglio conosciuto come legge comunitaria. A tale

11-*bis* per definire e trattare una materia che è di competenza della Commissione difesa. Si tratta di una

transito, trasferimento, trasbordo ed intermediazione dei prodotti per la difesa, e per il riordino dei procedimenti nella materia di cui alla che il Governo abbia voluto tentare di aggirare le normali procedure inserendo surrettiziamente una norma che non solo non può essere trattata in questo contesto,